non c'è nessuno

che, dai trapianti di cuore ai vaccini, alle sperimentazioni sulle forme tumorali e così via, hanno permesso di progredire

È altrettanto evidente che, nel contempo, è cresciuta una sensibilità a livello mondiale per rendere compatibile l'indispensabile ricerca - che deve continuare,

sanziona e indica, per ogni specie, come ci si deve muovere per garantire al massimo la protezione degli animali. Perché la discutiamo solo nel 2013? Perché da tre anni siamo fermi, in quanto in Italia non si vuole recepire la direttiva europea così com'è, ma si vuole fare di più; io dico: si vuole fare i primi della classe. Tant'è vero che anche nel provvedimento che discutiamo questa mattina, all'articolo 12, prevediamo tutta una serie di limiti, alcuni dei quali,

e noi scriviamo, all'articolo 12, che è proibita la ricerca sulle sostanze d'abuso condotta sui ratti. In Italia, quindi, non si potrebbe più fare ricerca riguardo la cocaina,

di organi) e l'applicazione sugli animali può consentire la creazione di un archivio di organi da trapiantare sugli uomini senza aspettare il decesso di una persona, per salvare milioni di vite umane.

per la farmacopea internazionale non è consentito brevettare un farmaco e metterlo in commercio se prima non è stato sperimentato su due tipi di animali, fra cui un primate. Dal momento che in Italia è stata chiusa una struttura

gli Stati membri non possono introdurre nel loro ordinamento criteri più restrittivi rispetto a quelli dettati dalla direttiva europea

quindi questa clausola di salvaguardia che impegna il Governo - lo ripeto per la seconda volta - ad applicare integralmente e a recepire totalmente tutti i criteri che la direttiva europea impone per salvaguardare e proteggere

dovessi scegliere se mettere a rischio la vita di un essere umano o quella di un animale, di un roditore, di un topo o di un cane, messo alle strette, sceglierei di salvaguardare la vita umana.

scrive e sostiene che, se allora il farmaco si fosse testato sulle cavie, 10.000 esseri umani non avrebbero dovuto sopportare per tutta la vita le conseguenze di questa mancanza di attenzione nei loro confronti. È un errore che storicamente è stato fatto. Dopo di che la comunità internazionale ha obbligato, prima di mettere in commercio un farmaco e di applicarlo sugli uomini, sulle donne e sui bambini, a testarlo sugli animali. È giusto che sia così. È giusto che questo venga fatto con tutte le cautele e le attenzioni del mondo, però credo che questo Senato debba avere ben presente che c'è una gerarchia dei valori e che prima dei roditori vengono gli esseri umani.

Cari colleghi senatori, oggi vi voglio guidare in una breve riflessione di tipo metodologico. Ormai l'Unione europea ha fagocitato l'attenzione normativa dei Paesi membri e l'Italia, dal momento che ha la vocazione di continuare a partecipare a questa unità continentale, vocazione che, a nostro parere, però, dovrebbe essere ratificata dal popolo per avere legittimità, deve ritrovare necessariamente un passo più giusto per stare dietro all'Europa. Sappiamo anche che il futuro svuoterà sempre di più i Parlamenti nazionali dal potere legislativo interno e lo delegherà alle rappresentanze in Europa, lasciando così ai nostri organi istituzionali - come già succede - un ruolo marginale che deve recuperare importanza attraverso una partecipazione attiva alla legislatura europea, e non passiva, come stiamo facendo. Ad oggi due leggi si sono succedute per rendere maggiormente organica la fase di formazione e recepimento della normativa europea, ma purtroppo - come dimostrano le decisioni di questi giorni - a livello operativo stiamo indietro anni luce. Questo è assolutamente inammissibile, com'è inammissibile che, a causa del lassismo della classe politica degli ultimi anni, il nostro Paese si trovi oggi ad inseguire l'attività normativa piuttosto che a parteciparvi attivamente. I precedenti Governi hanno solo approvato autodecapitazioni, come il MES e il *fiscal compact*, e hanno sostenuto con forza una moneta unica che non è solo una moneta, ma un metodo di governo che a noi non fa tutto questo bene e a causa della loro latitanza (perché siete stati tutti latitanti nelle normative europee) non hanno prodotto altro che un accumulo di procedure di infrazione (ad oggi più di cento), multe e direttive da dover passivamente recepire.

Tutte in due atti parlamentari: così, se si boccia il recepimento si bloccano tutte, con cifre astronomiche da pagare, cifre che il nostro Paese non può permettersi: questo è il solito ricatto sociale per far passare le cose in fretta. Noi siamo fermamente convinti, come Movimento 5 Stelle, che sia necessaria una rivisitazione della *governance* europea per porre al centro dell'attenzione e della procedura decisionale i cittadini. Quindi, dobbiamo prevedere la creazione di istituzioni che siano più rappresentative, perché queste non ci rappresentano affatto, con organismi votati dal popolo e quindi legittimati a prendere decisioni in nome e per conto del popolo, cosa che in questo momento non sta avvenendo. Il sistema normativo deve essere garantista di tutti i Paesi e consentire la partecipazione dei Parlamenti nazionali, ma non solo come collegi di indirizzo e di valutazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (questo a noi non basta), come veri e propri organismi che abbiano carattere vincolante per le politiche comunitarie. Il Parlamento europeo in questo modo verrebbe a trovarsi con sempre maggiori posizioni provenienti direttamente dai cittadini. Per noi nessuno deve rimanere indietro: questo è un motivo trainante del nostro movimento, e speriamo che lo diventi per tutti. E questo concetto non può prescindere da un percorso congiunto di confronto politico e democratico che sia garantista nei confronti di tutti i Paesi europei, con attenzione però alle diversità culturali (non possiamo essere omologati), storiche, territoriali e sociali, e soprattutto - cosa che non sta avvenendo - che persegua la protezione dai grandi potentati dalla speculazione economico-finanziaria.

in sede di prima applicazione della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, si compie un passo significativo nell'ambito del cambiamento del paradigma culturale e politico, che segna il passaggio dal mero adempimento degli obblighi

e coordinamento, ma anche maggior tempestività nell'adempimento degli obblighi europei, concretezza e capacità propositiva. Quell'Europa nata dai Trattati di Roma, con la scelta d'integrazione funzionalista, anche se progredita a tappe incerte, ci ha consegnato un patrimonio acquisito irreversibile, dall'elezione diretta del Parlamento europeo all'unione doganale, dal mercato unico alla libera circolazione di beni e servizi, all'Accordo di Schengen per il controllo delle frontiere esterne, alla cittadinanza europea e all'unità monetaria; e, sul versante istituzionale, dalla struttura a pilastri del Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona, che oggi, modificando il funzionamento delle istituzioni di un'Unione allargata a 28 Paesi membri, rende i meccanismi decisionali più efficaci con l'estensione della più democratici e trasparenti, perché più vicini ai Parlamenti nazionali. La legge italiana n. 234 del 2012 ne rappresenta lo strumento interno; strumento giuridico, ma che deve tendere al perseguimento degli obiettivi politici dell'Unione europea di medio e lungo periodo, quali quelli sanciti nel programma varato dalla Commissione per la strategia Europa 2020, per una crescita *smart*, intelligente perché basata sulla conoscenza, sostenibile perché in grado di promuovere l'economia verde, intelligente perché inclusiva, ovvero in grado di promuovere occupazione. Eppure questa Europa, nel periodo di crisi più difficile, ci è apparsa una cattiva madre, capace di imporre austerità e rigore nei conti pubblici e incapace di dare attuazione a quel principio di solidarietà che avrebbe dovuto accompagnare la cessione progressiva di sovranità degli Stati membri; vi è stata incapacità a condividere destini nazionali che diventano comunitari per prendersi carico, anche con fondi destinati, dei debiti nazionali e procedere a ristrutturazioni che non portassero vantaggio soltanto agli istituti bancari. A Roma l'azione del nostro Governo è riuscita a sancire il passaggio dai temi dell'Ecofin ai temi della disoccupazione giovanile, come riferito dal presidente Letta la scorsa settimana, rimettendo finalmente al centro della costruzione europea l'uomo, il cittadino europeo. Bisogna al rigore e la crescita, per un nuovo Patto di stabilità che agevoli gli investimenti degli enti locali, capaci di rilanciare l'economia; è necessario l'impegno a destinare i fondi strutturali e il Fondo sociale europeo, nello specifico, per sostenere l'occupazione giovanile. Quella della disoccupazione giovanile è una priorità e racchiude tutte le storture del nostro Paese. Ieri era l'Europa della generazione Erasmus; oggi è la fuga dei cervelli.

anche per violazione dei diritti dell'uomo; sono addirittura 600 le sentenze di condanna per i tempi troppo lunghi del nostro sistema giustizia. È proprio per questo continuo richiamo alle infrazioni che dobbiamo trovare la forza

per l'adeguamento agli obblighi europei. Un'ultima considerazione. In questo momento possiamo tranquillamente uscire da una posizione di sorvegliati speciali per diventare promotori veri e convinti del processo di unificazione europea.

questa Assemblea oggi deve delegare il nostro Governo a recepire alcune direttive europee e ad attuare altri atti dell'Unione europea. Tuttavia prendo spunto dal testo relativo alla trattazione di questi disegni di legge per spostare il punto di osservazione di voi colleghi su un argomento fortemente dibattuto in questo periodo. Mentre leggevo in questi giorni il provvedimento in esame e le materie presenti nel *corpus* delle direttive che ci apprestiamo a recepire, mi sono venute in mente le numerose discussioni, avvenute anche in questo consesso, circa l'opportunità che una sovrastruttura tentacolare e sovranazionale come l'Unione europea possa determinare, attraverso delle costruzioni formali e regolamentari di tipo generale, il vivere sostanziale di comunità di cittadini così distanti geograficamente, ma soprattutto distinti per storia, costumi sociali e microeconomie. Il dibattito pubblico su giornali, televisioni, radio, *web* ed ogni forma di informazione è tornato negli ultimi mesi di forte attualità, e non solo nel campo della comunicazione di massa ma, come ho avuto modo di appurare, anche nell'ambito accademico universitario. La crisi dell'economia dei Paesi mediterranei al cospetto della ricchezza sociale e dell'egemonia commerciale e finanziaria di quelli di etnia gallo-germanica, acuitasi in questi anni di primo monetarismo unitario, rischia seriamente di minare il raggiungimento agognato di un lungo periodo di *pax socialis*, che ci si aspettava di realizzare con l'attuazione della moneta unica. Fior di economisti e di pensatori contemporanei si stanno interrogando per cercare di capire se sia vantaggioso, per i Paesi che maggiormente hanno risentito della recessione, restare nel reticolato legislativo e regolamentare di Bruxelles o provvedere, secondo principi autonomistici, a sanare bilanci e configurazioni economiche nazionali. Lo scenario è diviso tra chi sostiene che è possibile sfidare gli Stati che dettano la linea della politica europea e chi ritiene che sia una follia porsi fuori dalle norme che noi stessi abbiamo concorso a produrre. Il problema giuridico finanziario non è di facile soluzione, o quanto meno è più insidioso di quanto potrebbe sembrare, in maniera forse troppo semplicistica. Quel che so è che molti imprenditori, nonché lavoratori e loro dipendenti con cui mi relaziono, sono spesso dell'avviso che i parametri imposti attraverso le direttive sono in alcuni casi deleteri al sistema produttivo

nel *mare magnum* di questi atti legislativi ci sono tante norme di buonsenso e consolidata sperimentazione pragmatica che ci spingono nella direzione del progresso sociale e del miglioramento della qualità della vita del nostro Paese. Per questa serie di motivi credo sia opportuno per noi includere e mettere a frutto le esperienze comunitarie contenute nel testo. Quindi esprimo con soddisfazione il mio voto favorevole alla delega al Governo per il recepimento di queste disposizioni e di questi atti nel nostro ordinamento.

Signor Presidente, ci ritroviamo un'altra volta con più di 30 direttive europee accorpate in soli due provvedimenti. Naturalmente sono tutte procedure di infrazione aperte, sono tutte procedure che ci costano soldi (o meglio, non costano a noi ma alla cittadinanza). Il Governo aveva promesso, all'atto del suo insediamento, che non avrebbe più fatto provvedimenti *omnibus*; si è dimenticato di aggiungere le parole «non altro che», nel senso che più correttamente si dovrebbe leggere «non faremo altro che provvedimenti *omnibus*». Per di più, queste direttive europee sono tutte finite in discussione nel giro di una decina di giorni, dopo essere state a fare muffa per due anni. eravamo in urgenza perché eravamo sotto infrazione; benissimo, però abbiamo aspettato due anni per poter dire che eravamo in infrazione. Forse questo sembra un metodo per far sì che poi le cose vengano discusse in poco tempo, in fretta e senza poter prendere decisioni ponderate e sensate. Pertanto vorremmo che si smettesse con questo metodo, possibilmente a partire dal prossimo atto legislativo; vedremo se questo potrà essere attuato. Tra l'altro, ancora una volta ci lamentiamo che l'Europa ci dica che dobbiamo fare certe cose, ma in realtà sono cose di assoluto buonsenso che avremmo dovuto fare da noi senza che qualcuno ce lo dicesse. Per esempio, non abbiamo bisogno che l'Unione europea ci dica che dovremmo certificare e controllare come vengono gestite le foreste e l'importazione di legname, perché negli ultimi anni abbiamo depauperato e distrutto le foreste della Romania (tanto per citare una Nazione che ha così tanta voglia di inguaiarsi con l'euro) sia come legname da opera che da costruzione, e persino come legna da ardere. Abbiamo importato sei milioni di tonnellate di legna da ardere dalla Romania, mentre abbiamo dei boschi che hanno continui schianti, come le abetine le abetine dell'Appennino (che, ricordiamo, sono artificiali, sono state impiantate dai monaci camaldolesi). Ebbene, nonostante questo, riusciamo ad andarci a prendere la legna all'estero, per non parlare di quello che facciamo quando importiamo la legna dall'Indonesia o dal Madagascar.

un insieme di falsità e di cose senza senso che veramente riempirebbero un vagone. Comunque vorrei dire brevemente che vi è in primo luogo, un fatto etico, nel senso che dovremmo cercare di avere un atteggiamento antispecista e quindi non privilegiare una specie animale rispetto alle altre. Non solo, ma l'attuale tecnica di calcolo ha permesso di simulare di simulare forse l'evento più complicato che si può verificare, cioè una detonazione nucleare, la quale - lo ricordiamo - avviene in qualche miliardesimo di secondo. Ebbene, la tecnica di calcolo è riuscita a simulare le incredibili quantità di collisioni neutroniche che avvengono nell'ambito di una detonazione nucleare, ed è possibile simulare in modo ottimale le dinamiche atmosferiche oppure il comportamento di molecole all'interno di un organismo. Nonostante questo, nonostante il fatto che più del 90 per cento delle medicine che hanno avuto successo nella sperimentazione animale poi sull'uomo non funzionino, si continua a parlare di sperimentazione animale. Qualcuno potrebbe dire che qui non si sta parlando di di fare o non fare sperimentazione animale: in realtà lo stiamo facendo, perché nel recepimento della direttiva europea stiamo comunque accettando la sperimentazione animale sotto forma ristretta. Se qualcuno veramente ritiene di essere contro la sperimentazione animale, cioè antispecista, dovrebbe dire: «Questa cosa non la accetto, perché non la posso accettare, dopo di che intervengo sulla legislazione nazionale e mi attivo in sede europea nella fase ascendente per dire che questa cosa in Italia non la vogliamo».

Come ho ribadito in Commissione ambiente, dove sono stato relatore del disegno di legge n. 588, è un fatto assolutamente positivo che il nostro Paese si adegui alle normative europee, scongiurando così il rischio di cadere in una procedura d'infrazione. Anch'io mi auguro davvero che sempre

è quello del venir meno di quel principio di sussidiarietà che deve restare come un valore assoluto, proprio per non tradire lo spirito originario dell'Unione europea, che pone tale principio tra quelli alla base della sua ragione di esistere. Questa è stata la motivazione alla base del mio parere positivo, condiviso a maggioranza dalla Commissione, sul disegno di legge n. 588, parere che in parte, devo dire, è stato stravolto da altre Commissioni: mi riferisco, in particolare all'articolo 27 (oggi diventato 26), modificato nella sostanza.

che si configura come strumento di attuazione bilaterale dell'Accordo di Madrid, che negli anni ha già ricevuto vari via libera sia da parte del Parlamento che del Consiglio dei ministri),

Pertanto, ad oggi manca solo l'ultimo passaggio, ovvero l'autorizzazione alla ratifica da parte del nostro Parlamento. La ratifica di questo accordo rappresenterebbe un fatto importantissimo in una visione dell'Unione europea come casa nella quale i popoli possono davvero crescere insieme. Solo per dare un'idea, cito dall'articolo 4 dell'accordo-quadro siglato tra Italia e Austria quali sarebbero alcune delle aree di costruzione sinergica: trasporti e comunicazioni, distribuzione dell'energia, tutela dell'ambiente, gestione di parchi transfrontalieri, artigianato, formazione professionale, sanità, cultura, sport, tempo libero, protezione civile, turismo, problemi dei lavoratori transfrontalieri in materia di trasporti, sicurezza sociale, posti di lavoro, disoccupazione. Sono tutti problemi che, data la contiguità sociale ed economica, meritano un approccio sinergico, al fine di generare un modello di crescita e di sviluppo nell'interesse di tutti, senza far venir meno le prerogative degli Stati di appartenenza dei vari territori interessati. Questo accordo rappresenta un valore aggiunto, un volano di relazioni, un passo importante verso quella democrazia dal basso che, da sola, può costruire l'Europa dei popoli e delle regioni, che tutti vogliamo, ma che facciamo fatica ad accettare; eppure è l'unica Europa che può reggere, se non vogliamo che l'Unione fallisca sotto il peso dei diversi nazionalismi I nostri tre territori hanno costituito il GECT (Gruppo europeo di cooperazione territoriale): è il secondo in Italia e il ventunesimo in Europa e sta funzionando davvero bene. Il GECT rappresenta oggi l'unica strada giuridicamente percorribile, ma il protocollo aggiuntivo aprirebbe scenari importanti e strategici anche per altre regioni di confine: pensiamo a quelle che si affacciano sui Balcani, ora che la Croazia è entrata a tutti gli effetti nell'Unione europea. So che su questo ordine del giorno vi sono problemi di improponibilità, e attendo la pronuncia della Presidenza; se non dovesse essere accettato, mi faccio però carico fin d'ora di presentare un disegno di legge che, mi auguro, questo Senato vorrà approvare. L'Italia non può più reggere questa contraddizione:

il Parlamento e il Governo vogliano quanto prima procedere con la ratifica, sempre con l'idea che tutto questo vada nella direzione auspicata, cioè quella di una politica che rende libera la società e la mette nelle condizioni di poter esprimere tutte le proprie potenzialità, l'unico modo per uscire concretamente ed efficacemente dalla crisi. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, siamo consapevoli dell'importanza strategica di questa discussione, perché la legge comunitaria, ora sostituita dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, deve rappresentare un'occasione preziosa per fare il punto sulle modalità di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione, e soprattutto sugli effetti di tale partecipazione. Infatti, dal canto suo, la Commissione europea esprime doglianze nei confronti di alcuni Stati, nella fattispecie l'Italia, per la mancata, parziale o errata applicazione delle disposizioni della legislazione europea: di qui, la necessità di correggere eventuali inadempienze per recepire correttamente le disposizioni. D'altro canto, però, leggendo entrambi i disegni di legge in discussione, si trova ripetuta numerose volte la parola «obblighi». legittimo a questo punto un dubbio, perché forse si è superato qualche limite: dobbiamo chiederci se l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea non stia calpestando le prerogative degli Stati e dei suoi cittadini. Il sospetto è molto forte, e questo rischio lo si corre nel momento in cui il Governo e il Parlamento si adeguano a decisioni prese in Europa che non tengono conto delle specificità e delle peculiarità del nostro Paese; specificità che non possono essere comprese da chi è lontano e ragiona in termini astratti su realtà che non conosce e non vive quotidianamente. È il caso dell'articolo 33, prima articolo 35 della legge europea, che pretende dall'Italia l'immediata restituzione del 100 per cento di tasse e contributi sospesi alle imprese colpite dai sismi del 1997, del 2002 e, in ultimo, da quello aquilano del 2009,

perché se l'Europa non ha voluto guardare alle difficoltà evidenti in cui si sono trovate ad operare ed operano tuttora le nostre imprese, in parte, forse, la responsabilità è stata anche nostra; nostra; evidentemente non abbiamo fatto sentire a sufficienza la nostra voce e non abbiamo avuto il coraggio di assumere posizioni incisive e, soprattutto, non siano stati presenti nelle fasi e nelle sedi in cui le misure sono state adottate. Dobbiamo invece avere coraggio nel far valere le ragioni dell'Italia. Nel caso delle imprese, e parlo soprattutto per quelle dell'Aquila, la motivazione che

e sono state svantaggiate a prescindere dal livello di danno subito. Pertanto, l'intervento dello Stato non ha avuto altro effetto che quello di ripristinare una parità di condizione tra imprese operanti in queste situazioni di calamità e imprese limitrofe. Quindi, in nome del rispetto degli obblighi comunitari, le istituzioni italiane penalizzerebbero imprese già messe a dura prova da da questi eventi naturali così disastrosi. Penso quindi che in questo momento debba entrare in gioco il buonsenso; un buonsenso che deve entrare in gioco anche in tante altre occasioni. Voglio riportare un altro esempio di una direttiva che non è

Le concessioni demaniali infatti potrebbero essere messe a bando pubblico e, quindi, passare attraverso la vendita all'asta, nonostante la specificità italiana che rende le nostre coste e la loro organizzazione uniche al mondo. In Italia proprio gli automatismi nel rinnovo delle concessioni hanno permesso un grande sviluppo e imprese medio-piccole, quando non a carattere familiare, hanno raggiunto risultati inimmaginabili, contribuendo in maniera decisiva all'economia nazionale. Perché 27 Stati, seduti attorno ad un tavolo, devono avere il diritto di decidere dell'utilizzo delle spiagge di soli tre Stati che hanno le coste balneabili? Il sospetto è che entrino in gioco anche altri interessi ed altre logiche. E non mi sorprenderebbe se proprio da quegli Stati, privi di spiagge balneabili, partissero flussi di capitali e di imprenditori desiderosi di investire sulle nostre spiagge, in nome della sbandierata libertà di concorrenza. Per questo credo che proprio l'utilizzo del buon senso imponga, anche su questo tema, una riflessione. Pertanto, da un lato, chiediamo al nostro Governo di svolgere un'azione maggiormente incisiva in sede europea, d'altro, però, dobbiamo usare bene la discrezionalità che ci è riconosciuta nelle modalità di recepimento delle norme comunitarie. Infatti, decisioni assunte a maggioranza da un'entità - l'Unione europea astratta e lontana possono provocare ripercussioni gravi sulle specificità nazionali. Proprio per questo, gli Stati membri dispongono di quel margine di discrezionalità, e mi auguro che in Italia si inizi a farne buon uso.

«L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto»: ho citato Robert Schuman, un padre dell'Unione europea, tanto stimato e caro anche a De Gasperi. Questo si può fare mediante la realizzazione di un punto di incontro, dove queste esperienze si confrontano e si selezionano, così dando vita a nuove forme di comunità ispirate ad una più grande libertà e ad una più giusta vita sociale. L'Unione europea è il nostro punto di incontro; le normative europee sono il risultato del confronto e della selezione degli ideali e dei valori: questo dovrebbe essere. Leggo dalla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che l'azione del nostro Paese in materia di occupazione e politiche sociali ha come obiettivo prioritario il potenziamento dei regimi di protezione sociale e delle politiche di attivazione, sostegno e promozione dell'inclusione sociale e dei mezzi di sostentamento adeguati, in attuazione della strategia Europa 2020, secondo il programma della Commissione 2013. Orbene, la strategia Europa 2020, tra l'altro, si prefigge l'obiettivo di

queste persone costituiscono il maggior peso sociale, in quanto sono totalmente dipendenti dal nostro sistema di sicurezza sociale. Inoltre, sono più di 9 milioni i cittadini italiani che non percepiscono alcun reddito e - quindi - a rischio di povertà e di esclusione sociale. Il Movimento 5 Stelle ritiene che bisogna operare una complessa razionalizzazione ed una semplificazione degli strumenti di sostegno al reddito attualmente esistenti, al fine di pervenire, al pari degli altri Paesi europei, all'introduzione del reddito di cittadinanza

card*, invece di soffermarsi su tale strumento, che deve essere inteso non disconnesso da una ristrutturazione del sistema dei servizi per l'impiego.

parliamo spesso di competitività del sistema industriale italiano e della necessità di legare questa competitività all'innovazione e alla ricerca.

l'Italia entri nella procedura di collaborazione rafforzata quanto al brevetto unico europeo. Il brevetto, come sapete, è il documento che cristallizza i risultati ottenuti nel campo della ricerca applicata da chi lo deposita, cioè le imprese, e costituisce uno dei principali elementi di competitività per chi lo raggiunge. Il sistema italiano della media, piccola e anche della grande impresa non è all'avanguardia da questo punto di vista, anche perché è rimasto legato per troppo tempo ad una visione ristretta di questa funzione cruciale nello sviluppo delle imprese. Legare semplicemente alla dimensione nazionale, come si è fatto finora, la costruzione dei brevetti e poi la successiva estensione nei diversi Paesi apparentemente costituisce una limitazione di costi: il brevetto nazionale, infatti, richiede un investimento di ratifica inferiore a quello europeo ma poi,

almeno 40.000 euro per brevetto). Se invece aderiamo al brevetto europeo, tali costi si abbassano fra i Certo, sono un po' più alti di quelli che si rendono indispensabili per la mera dimensione nazionale. Qui però dobbiamo decidere se per difendere situazioni di arretratezza del nostro sistema vogliamo impedire a chi lo voglia di aderire

che rivestono un'importanza rilevante anche per la vastità dei temi trattati, che hanno una ricaduta pratica, diretta, su molti ambienti delle nostre amministrazioni. A questo proposito vorrei svolgere solo una breve considerazione, che ho già condiviso con i colleghi della Commissione igiene e sanità, riguardo agli effetti che le normative europee hanno in particolare sui territori di montagna.

i regolamenti mettano in seria difficoltà alcuni settori lavorativi, come quelli degli agricoltori e degli allevatori di montagna, o dei produttori primari,

pensate probabilmente per le pianure dell'Olanda, della Francia, della Germania, ma con scarsa considerazione dei territori montani. Questo si traduce nell'impossibilità per le Regioni e lo Stato stesso di apportare modifiche adeguate, con possibili ricadute in termini di sanzioni dell'ordine di migliaia di euro ad aziende agricole e montane che si trovano già in difficoltà oggettiva, per le quali queste multe rappresentano a volte la classica goccia che fa traboccare il vaso di una vita sempre più difficile, piena di controlli di tutti i tipi e di burocrazia. quindi, signor Ministro, di lasciarle questa sollecitazione a farsi carico di tali criticità e a trasmetterle alle autorità europee e agli eletti nel Parlamento europeo,

corretto il ritardo con il quale il Parlamento è arrivato all'esame di questi provvedimenti

esame sono stati affrontati con un'ottica giusta: l'impostazione data dalla Commissione è quella di una nuova responsabilità rispetto agli obblighi

a definire e a confezionare provvedimenti, in qualche parte modificativi delle direttive e dei regolamenti oggetto dell'azione di recepimento del Parlamento, che mantengono

le infrazioni riguardino settori particolarmente sensibili, come l'ambiente, le politiche sociali, le attività di inclusione, i diritti umani. infatti più distrazione per tali questioni, che attengono alla vita di tutti noi - l'economia, la fiscalità - piuttosto che per altre vicende che riguardano alcuni in particolare. Inoltre, signor Presidente, mi pare sia giusto e doveroso aprire una questione sulla applicabilità dell'articolo 81 della Costituzione in queste circostanze. Infatti, vi è una prassi, un orientamento che ritengo ormai inaccettabile, per cui ogni adattamento del funzionamento della pubblica amministrazione alle nuove disposizioni comporta oneri e viene applicato quasi automaticamente l'articolo 81 della Costituzione come un diniego ad introdurre quelle innovazioni. Così, abbiamo un sistema pubblico particolarmente rigido che trova una forza conservatrice ulteriore nella interpretazione per cui ogni modifica di natura procedurale alla quale siamo costretti

il nostro destino, ripetendo frasi come: «dobbiamo diventare più europei», «noi siamo all'avanguardia di questo movimento», «noi vogliamo costruire finalmente un'Unione europea in cui la nostra partecipazione sia attiva e determinante».

comporti effettivamente un onere aggiuntivo per poter porre il veto che discende dall'articolo 81 della Costituzione. Infine, mi sembra

pagavamo un ritardo colpevole, siamo riusciti ad andare avanti in modo totalmente condiviso senza registrare alcuna divisione significativa all'interno della Commissione.

la lettura della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 solleva non poche perplessità. La relazione ci parla di un percorso già segnato di progressiva integrazione economica e riforma strutturale, termine funesto come vedremo più avanti, dell'economia italiana come se non esistessero scelte da compiere e ponderare, decisioni su cui riflettere, scenari da indagare, questioni da approfondire. La relazione vorrebbe farci credere che viviamo nel migliore dei mondi possibili, che l'Unione europea non conosce criticità, se non quelle esterne ed esogene, quale una crisi economica vissuta come *shock* esterno o al più addebitata a una generica globalizzazione. Celebra la gloria e i fasti di una politica di integrazione apparentemente priva di ombre, come se nessun errore fosse stato fatto, come se a nulla bisognasse rimediare. Mai, se non retoricamente, viene annunciato o invocato il costituirsi di momenti di riflessione e confronto sul percorso fin qui svolto, sulle scelte fatte, sulla legittimità e democraticità dei meccanismi di governo del mercato unico e della moneta unica, sulla possibilità di una partecipazione maggiore dei popoli europei alle decisioni che calano dall'alto. Più che una relazione programmatica, questa appare un panegirico sulle politiche europee, come quando viene celebrato lo strabiliante successo dei parametri di Maastricht e dell'unificazione monetaria e di mercato, là dove la relazione afferma, cito testualmente: «Dopo il 1992, la realizzazione delle "quattro libertà" (libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali) ha dispiegato un enorme potenziale di crescita e dato avvio a un importante processo di sviluppo economico e sociale». Questa affermazione ci fa sorridere, se consideriamo che l'ultimo ventennio è stato quello a più bassa crescita dal Dopoguerra, e che gli ultimi anni hanno visto dispiegarsi una depressione economica persino peggiore, per l'Italia, di quella del 1929. Ma c'è un altro aspetto di questo passaggio che ci preme sottolineare: l'enfasi sulle quattro libertà supposte a fondamento della futura, ipotetica prosperità dei popoli europei. Perché per il Movimento 5 Stelle il porre a fondamento del progetto europeo quattro libertà, che corrispondono indistintamente a cittadini, merci, servizi e capitali, va in rotta di collisione con la Costituzione repubblicana, che non equipara cittadini, merci, servizi e capitali nella titolarità di diritti o libertà, ma anzi anzi subordina la libertà economica al conseguimento di fini sociali (articolo 41 della Costituzione). Come sempre più osservatori rilevano, l'eccessiva enfasi posta dall'Unione europea sulla dimensione economica, a volte anche a scapito della dimensione dei diritti e della legittimità democratica, è uno dei problemi del nostro tempo ed esige in quanto tale analisi e decisioni all'altezza del momento, non peana autocelebrativi indossando i paraocchi. La depressione che attanaglia l'Europa mediterranea, in particolare, e che nel volgere di pochi anni ha comportato anche una crisi politica, sociale, in alcuni Paesi (come la Grecia) addirittura umanitaria, ci impone di rivedere alcuni presupposti e scelte. Ci impone di fermarci per riflettere. Allora proviamo a riflettere su alcuni snodi centrali del documento. Il Governo si impegna circa «la prosecuzione di un consolidamento fiscale favorevole alla crescita», il che è un evidente ossimoro. Il consolidamento fiscale, comprimendo la spesa pubblica e la domanda interna, può avere come unico esito la la contrazione dell'economia e non certo la crescita. Questo ormai lo sanno anche i bambini, ma il Governo prosegue imperterrito nella sua opera di mistificazione dei principi basilari dell'economia. Il Governo promette fedeltà ai trattati europei che impongono le misure di austerità. Ammesso e non concesso che l'ossimoro rigore-crescita sia realizzabile, lo strumento con cui si intende perseguire questo obiettivo, cioè la fedeltà ai trattati dell'austerità, confligge evidentemente con un altro obiettivo programmatico dichiarato nella relazione, cioè del "coordinamento macroeconomico". Affidare il coordinamento macroeconomico al *fiscal compact* e al *growth and jobs compact* costituisce un'altra contraddizione in termini. Il *growth compact* e i trattati in cui si in cui si articolano impongono indiscriminatamente misure di rigore e austerità a tutti i Paesi membri, indipendentemente dalle rispettive posizioni riguardo alla bilancia dei pagamenti, al ciclo economico, all'indebitamento estero. Un reale coordinamento macroeconomico nell'eurozona - ce lo dicono i *report* della *United Nations Conference on Trade and Development*, ma potrei anche citare i rapporti di altri istituti, quali ad esempio il *Working Paper*

stimolino la loro domanda interna con manovre espansive, offrendo ai Paesi in *deficit* la possibilità di aumentare le loro esportazioni per recuperare il *gap* di competitività. I differenziali di competitività, inoltre, sarebbero attenuati dall'aumento dell'inflazione nei Paesi in *surplus* commerciale conseguenti alle manovre espansive. Sappiamo, però, quale terrore la parola inflazione, seppur controllata, generi nel popolo tedesco. Tutto questo non è previsto nel *growth compact*, che ignora le differenze fra i Paesi in *surplus* e in *deficit* commerciale, così come come le differenze fra Paesi creditori e debitori. Imponendo una disciplina fiscale uniforme e indifferente al ciclo economico, il *growth compact* di fatto nega il coordinamento delle politiche macroeconomiche previsto dai trattati fondativi dell'Unione europea (in particolare, l'articolo 5 del regolamento

Veniamo, allora, a discutere della partecipazione dell'Italia all'Unione monetaria, tema, anche questo, trattato in modo acritico e apologetico nella relazione. Per superare questa cortina propagandistica vale la pena leggere i *report* della Commissione europea (mi riferisco all'esame approfondito per l'Italia del 30 maggio 2012) che sostengono come dall'introduzione dell'euro - cito testualmente - «la perdita di competitività sui costi è uno dei fattori principali alla base del declino della bilancia commerciale dell'Italia» «L'andamento del tasso di cambio effettivo reale fa pensare all'instaurarsi di un divario competitivo (...) fra l'Italia e altri Paesi della zona euro». La Commissione stima una sopravvalutazione del cambio nominale rispetto al cambio reale pari al 10 per cento rispetto agli altri Paesi europei e del 25 per cento rispetto alla Germania. Se il cambio nominale dell'euro è troppo forte per l'Italia, per la Germania invece è troppo debole, favorendone le esportazioni a danno dei suoi *partner* commerciali, cosa che peraltro pone un ulteriore ostacolo al coordinamento delle economie fra Paesi membri di fronte all'indisponibilità della Germania ad affrontare tali squilibri (aspettiamo fiduciosi le prossime elezioni tedesche). Il combinato della sopravvalutazione dell'euro rispetto al tasso di cambio reale italiano con la sottovalutazione dell'euro rispetto al tasso di cambio reale della Germania (nostro principale *partner* commerciale) costituisce, al contempo, un volano per l'economia tedesca e un macigno inaggirabile per il sistema industriale italiano. La tara sui costi di produzione grava non solo sull'*export,* ma anche sul mercato interno, invaso da merci e servizi di Paesi concorrenti (*in primis* la Germania stessa) che godono di un tasso di cambio nominale debole e di un divario competitivo cumulato negli anni che non potrà che aumentare progressivamente. Un tale *gap* nei costi di produzione è pressoché irrisolvibile allo stato attuale delle politiche europee, ed è inutile a tal riguardo vaneggiare parlando di ricerca, innovazione, flessibilità, sburocratizzazione, parole tanto care al «modello unico» che ci governa e sicuramente utili in tempi di crescita, mentre si rivelano impotenti durante una spirale depressiva, come quella attuale, come strumenti per affrontare quello che la stessa Commissione europea definisce il divario nei costi di produzione Insomma, offrite aspirine per curare una pestilenza! La fissità del cambio, in assenza di un coordinamento macroeconomico fra *partner* commerciali, produce un divario di competitività che si cumula e amplia ogni anno che passa, strangolando l'economia italiana in una spirale di cui non si vede la fine. Il modello unico non vuole affrontare l'argomento di fronte all'opinione pubblica, preferendo lasciar morire l'economia italiana tramite una lenta ma inesorabile eutanasia. La relazione oggi in esame nemmeno nomina questa criticità nel vano tentativo di ignorare l'elefante nella cristalleria, cristalleria, avendo pure il coraggio di affermare che il Governo si sarebbe speso - cito testualmente - per «un'equa condivisione dei benefici e dei rischi della moneta unica». Se questa è equità forse dovremmo iniziare a non parlare più di integrazione europea, ma di annessione all'Europa.

delle lacerazioni profonde, che portarono all'immobilismo e comunque alla chiusura rispetto a queste migliorie in Senato, mentre, grazie all'impegno di tutti, alla Camera dei deputati si ottenne un esito favorevole (sono certa

di cani, gatti e primati, mentre ovviamente nessuno è in grado di intervenire, o comunque nessuno vuole ostacolare la ricerca e la sperimentazione che, purtroppo, viene ancora fatta su altri animali. Adesso le cose sono cambiate, anche se potrebbero essere migliorate. In qualche modo, in questo nuovo Parlamento, riproponiamo una norma che, grazie al lavoro svolto in 14a Commissione, grazie al lavoro del presidente Chiti, dei relatori

accettabile sul filo di quello che è il ragionamento etico e morale che ognuno di noi pone quando parla di ricerca e quando parla comunque della vita di un altro essere vivente.

L'Italia è spesso incorsa in infrazioni pesanti, milioni di euro che gravano sulle tasche dei cittadini, proprio per la mancata tutela degli animali. Penso all'ultima infrazione, che ci è stata comminata nel 2010, relativa direttiva sugli uccelli e in particolare i piccoli migratori, uccellini dai 20 ai 40 grammi di peso che migrano dai Paesi nordici dell'Europa, arrivano dalla Scandinavia e dalla Finlandia, e dopo aver percorso migliaia e migliaia di chilometri, a causa delle deroghe regionali,

purtroppo nel nostro Paese è ancora più comodo ed è ancora più facile massacrare animali per gli esperimenti, far procedere comunque la ricerca sulle basi dell'ordinarietà, piuttosto che investire denaro, scommettere e mettersi alla prova con i metodi alternativi, investendo soldi e cervelli. È più comodo e più facile comprare un cane o un gatto, usarlo il più possibile e poi, con una pietosa, ma anche ipocrita, anestesia o comunque eutanasia, metterlo a riposo. Costa di più più investire nei metodi alternativi, ma è quello che ci chiede di fare la ricerca internazionale. Ciò comunque non è escluso, perché nel testo concordato dell'articolo 12 viene mantenuta la possibilità di sperimentazione per tutta l'alta ricerca.

e meglio senza intervenire troppo sul bilancio pubblico. Noi siamo stati più volte condannati, ad esempio, sulla direttiva relativa alle galline ovaiole: le multe sono troppo basse, e quindi anche gli allevatori preferiscono pagare - se la pagano - una piccola multa, piuttosto che comprare una

Anche perché siamo tutti teoricamente già preparati quando i provvedimenti arrivano in Aula. Quindi non starò a ripetere delle cose che già dovremmo conoscere. Faccio solo due brevissime considerazioni di carattere generale: la prima sulla tecnica e - se mi consente - addirittura la «tecnologia» normativa che sta alla base di questi provvedimenti; la seconda sulle ricadute di questi provvedimenti sul sistema normativo complessivo. Sul primo punto, sul progresso che chiamerei tecnico della legge, sappiamo che stiamo davanti alla prima legge di delegazione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012, in attuazione del Trattato di Lisbona. Si tratta di un strumento normativo molto avanzato anche rispetto a molti altri Paesi europei, per cui forse ogni tanto possiamo anche essere contenti dei progressi che facciamo. Dopo le leggi La Pergola e Buttiglione degli anni scorsi, siamo davanti ad un salto di qualità importante dello strumento normativo. Sono in qualche modo lontani i tempi in cui l'Italia era sempre l'ultima ruota del carro nell'attuazione delle direttive comunitarie. Abbiamo una chiara separazione tra la fase ascendente e la fase discendente, con due leggi separate e diverse. La prima chiaramente è più importante per il ruolo che attribuisce al Parlamento; la seconda è meno importante, perché si tratta di obblighi che ‑ mi piace ricordare in gran parte spetterebbero alle Regioni, se sapessero fare adeguatamente e sempre il loro lavoro di dare attuazione alla normativa comunitaria nelle materie di loro competenza. Quindi, va riconosciuto che abbiamo finalmente uno strumento adeguato; la speranza è che il Parlamento familiarizzi al meglio con questa nuova secondo punto (quali conseguenze avranno cioè questi provvedimenti sul sistema complessivo), si tratta di leggi prevalentemente tecniche che servono, soprattutto la legge europea, ad arginare delle procedure di infrazione e a recepire la giurisprudenza della Corte di giustizia e le direttive europee. Ma l'ambito delle materie coperte è vastissimo e soprattutto riguarda un insieme eterogeneo di materie, che rendono più efficace il godimento delle libertà stabilite dal Trattato, in particolare l'accesso alle professioni, il riconoscimento dei servizi svolti all'estero, il diritto di soggiorno, l'accesso di alcune categorie di stranieri alla pubblica amministrazione. Sono dei provvedimenti di cui magari si parla si parla poco, ma che aprono realmente e finalmente il nostro Paese al pieno godimento delle libertà dei trattati, volenti o nolenti, perché molti sono frutto di procedure di infrazione. con questo percorso si avvia a diventare effettivamente più europea. Si vede che siamo soltanto all'inizio della sperimentazione di questo strumento legislativo, perché la legge copre circa soltanto un quarto delle procedure di infrazione attualmente aperte nei confronti dell'Italia. Ma certamente dobbiamo guardarlo come un primo importante passo, e l'auspicio è che la prossima legge europea sia meno occupata con le procedure di infrazione e più con il potenziale che queste leggi hanno, per consentire un vero progresso di tecnologia normativa, su cui queste leggi si fondano, che può portare il nostro Paese finalmente all'avanguardia in Europa, almeno in questo campo. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il disegno di legge in esame è figlio di una importante riforma che pone al centro un nuovo modo di dialogo fra Governo e Parlamento: più partecipazione del Parlamento alla fase di formazione delle normative e delle politiche europee e maggiore rapidità nell'attuazione delle direttive stesse.

legge comunitaria, principale strumento di attuazione della normativa europea, si sdoppia in legge di delegazione europea e in legge europea. All'origine di tale sdoppiamento c'è la consapevolezza che il precedente impianto presentava aspetti problematici, una sorta di abuso dello strumento stesso, che tendeva a farlo diventare una sorta di legge *omnibus*. Con questo sdoppiamento i ritardi dovrebbero essere superati, garantendo un *iter* più snello e veloce. È previsto che la legge di delegazione europea contenga solo le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive e delle decisioni da recepire nel nostro ordinamento, mentre la legge comunitaria tutti gli atti volti alle relazioni esterne dell'Unione. Entrando nel merito della legge di delegazione europea, per quanto riguarda il campo sanitario troviamo deleghe di grande interesse nel campo della medicina transfrontaliera. Chi è in Commissione sanità questo è quasi un mio pallino, ma temo fortemente che se non apriamo un dibattito e una riflessione ponderata su tale argomento potremo avere notevoli problemi. Tale direttiva disciplina i diritti dei pazienti all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente nell'ambito dell'Europa oggi a 28. Questa delega aprirà un grande dibattito e, pur riconoscendo l'assoluta bontà del provvedimento, si dovrà ponderare molto bene i meccanismi di rimborso delle prestazioni

sull'impatto che avrà sul nostro Servizio sanitario nazionale e regionale, in modo particolare per le Regioni confinanti con altri Paesi europei. Altra delega estremamente importante è la direttiva sulla farmacovigilanza. Lo Stato potrà, con azione urgente, sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio e vietare l'uso del medicinale per tutelare la salute pubblica. In questo campo noi siamo certamente i primi in Europa. La nostra rapidità di valutazione e di eliminazione dal commercio di un farmaco che può nuocere alla salute pubblica non ha pari in Europa, e di questo dobbiamo essere molto orgogliosi. Tralascio altri aspetti contenuti nel provvedimento per concentrarmi su una annosa questione: la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Il mancato recepimento entro il termine del 10 novembre 2012 ha indotto la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione per la mancata adozione delle misure di attuazione che garantiscono l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva del 2010 sulla protezione

ritengo che la 14ª Commissione abbia trovato un'ottima soluzione e sintesi con il comma 2 dell'articolo 12 che desidero leggere, perché esso ci mette al riparo da tutto: «Nell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali». Questo è un giusto approccio che ci inserisce a pieno titolo all'interno delle ricerche e delle protezioni europee, e soprattutto non farà fuggire i finanziamenti in materia di ricerche che si svolgono nel nostro territorio. Su questo abbiamo assistito negli ultimi anni ad una guerra senza confini che ha fatto impallidire la diatriba tra guelfi e ghibellini. Speriamo di segnare, con questo provvedimento, uno stop, una tregua. Ne abbiamo assolutamente bisogno. Per quanto riguarda la legge europea 2013, abbiamo una lunga serie di procedure di infrazione da sanare e di casi di EU Pilot che mirano a garantire risposte più rapide e complete riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione europea, in particolare quelle rivolte da cittadini o imprese. Nello specifico ci sono pronuncie in materia di società fra avvocati, monitoraggio fiscale, affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Termino, signor Presidente, signor Ministro, affermando che questo nuovo modo di trattare le direttive comunitarie deve vedere sempre più la partecipazione del Parlamento, perché sappiamo bene che sulla base del recepimento delle direttive europee negli ultimi anni è cambiata molto anche la politica italiana. Si dice sempre che l'80 per cento delle nostre leggi deriva da direttive europee. Pertanto, non possiamo stupirci quando viene adottata qualche direttiva che non ci piace, facendo finta che ci cada sulla testa, se non operiamo da subito sulla formazione delle direttive stesse. Questo nuovo modo di operare fa sì che il nostro Parlamento sia sempre più coinvolto nelle scelte che il Paese deve compiere in Europa e aumenta la trasparenza delle scelte. Pertanto, signor Ministro, salutiamo con favore questo tassello che certamente aumenterà la legittimità democratica dell'azione del nostro Paese verso l'Europa. *(Applausi

una modifica importante delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, prevedendo - credo correttamente - lo sdoppiamento della legge comunitaria in due provvedimenti, ossia la legge la legge europea, che contiene le disposizioni rivolte all'adeguamento, e la legge di delegazione per il recepimento. Per la prima volta

nel rapporto dello Stato italiano con la legislazione europea, anche perché ci troviamo in una situazione non certamente brillante in rapporto

il Governo attuale - sono stati certamente molto rigidi nel recepire e applicare in modo anche pedissequo gli impegni (penso, per esempio, a tutte le questioni che riguardano il *fiscal compact*), ma non sono invece altrettanto rigidi nell'integrare

essere parte dirigente nell'integrazione europea, nel costruire l'unione dei popoli, nel costruire la forte unità politica dell'Europa, mentre siamo tra i Paesi che maggiori ritardi rispetto all'adeguamento alla legislazione europea. È evidente che può capitare che ci siano dei contrasti tra gli interessi del nostro Paese e l'Europa, ma questo deve precedere il momento dell'adozione della direttiva, e spesso - lo dico anche al

discusso e votato il decreto sull'efficienza energetica, che riguardava anche il recepimento della direttiva, e anche lì con ritardo. Ritardo significa che, dal punto di vista degli obiettivi 20-20-20, certamente ci stiamo posizionando, ma potevamo essere parte dirigente di un processo molto virtuoso, anche dal punto di vista dei benefici

perché si è tentato di fare un lavoro importante, un lavoro che ha tentato, sia sul fronte della legge europea che su quello delle la legge di delegazione europea europea di fare dei passi avanti. In particolare, io mi voglio soffermare sui risultati, certamente importanti, che sono stati conseguiti per quanto riguarda, ad esempio, il recepimento della direttiva sulla vivisezione, la cosiddetta protezione degli animali. Certamente non è quello che, personalmente, molti di noi in quest'Aula avrebbero voluto (noi pensiamo che l'utilizzo degli animali nella sperimentazione non solo non faccia bene agli animali, ma non giovi né alla ricerca né agli agli umani), ma non possiamo non riconoscere, e di questo ringraziamo chi ha collaborato, dei significativi passi avanti nel recepimento della direttiva. Lo voglio dire: potrebbe essere la prima volta (e non capita frequentemente) che l'Italia possa essere un Paese guida, anche per gli altri Paesi europei. Infatti, le norme, che speriamo quest'Aula approvi, sono norme tali da permettere di essere un punto di riferimento avanzato: e lo voglio dire qui. È chiaro che si tratta anche di una battaglia culturale, di un passaggio culturale che noi dobbiamo compiere per superare quell'antropocentrismo

persone. Ricordiamolo sempre, perché il benessere della specie umana è legato alla capacità di essere in armonia con gli altri esseri viventi. Se il Senato riuscirà a compiere questo passo in avanti, sarà davvero un momento importante, che potrà dare segnali significativi per una ricerca e una scienza che davvero

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la prima volta il Parlamento è chiamato ad esaminare il disegno di legge per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti di Unione europea secondo le nuove

particolare importanza, alla luce della mancata approvazione delle due leggi comunitarie per il 2011 e il 2012 e, naturalmente, alla luce dei ritardi conseguenti dell'Italia nell'esecuzione dei suoi obblighi di componente dell'Unione. Ricordo, come sottolinea la relazione tecnica del provvedimento, che, in caso di mancato o erroneo recepimento degli obblighi europei, le sanzioni si articolano in due voci: una penalità, penalità, che va da 10.000 euro fino 600.000, per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza di condanna del tribunale di prima istanza della Corte di giustizia europea; una somma forfettaria di oltre otto milioni di euro che sanziona la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza e la seconda della Corte di giustizia, a norma dell'articolo 260 del I relatori hanno illustrato gli articoli sui quali si è concentrata la discussione in Commissione, e sui quali torneremo più tardi. Vorrei ora soffermarmi su una considerazione politica di fondo circa la partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Ieri è stata una bella giornata per gli italiani: il fatto che Barroso abbia annunciato l'uscita dalla procedura di *deficit* e promesso una maggiore flessibilità per i prossimi bilanci

Tutti insieme abbiamo evitato un clamoroso, ma annunciato crollo economico e abbiamo ripreso in mano il nostro destino. Bisogna riconoscere che il presidente Napolitano e il presidente Monti hanno saputo traghettare il Paese superando numerosi ed insidiosi scogli; oggi tocca al Governo Letta e alla sua maggioranza non sprecare l'occasione di poter fare investimenti strategici per la crescita, rimanendo nei parametri europei. Scelta Civica per l'Italia s'impegnerà affinché questo avvenga. Schroeder ha detto che le riforme strutturali possono funzionare solo congiuntamente ad una traiettoria di crescita. Sappiamo tutti che le azioni per la crescita con il necessario respiro si possono impostare e mettere in moto soltanto a livello europeo, rafforzando e spingendo più avanti i processi d'integrazione che proprio con la crisi hanno iniziato a prendere corpo. Infatti, a risultati del genere non si arriva, come abbiamo sperimentato in questi anni, mantenendo immutata una *governance* fortemente intergovernativa come quella attuale. Persino il presidente francese Hollande sembra finalmente essersene accorto e pare voler abbandonare l'Europa delle Patrie dei suoi predecessori per mettere la Francia sulla strada dell'integrazione sovranazionale. come ha osservato qualche tempo fa Giuliano Amato, saremmo noi inadeguati a capire le ragioni degli altri, se non ci rendessimo conto che gli altri sanno leggere di noi non soltanto l'entità del debito,

gli andamenti ciclici si sovrappongono a gravi debolezze strutturali ben anteriori alla stessa crisi. Mi limito a fare un esempio: si stanzia troppo poco per l'edilizia scolastica. Il ministro Carrozza poco tempo fa

Perché di quei pochi milioni stanziati dal CIPE tre anni fa neppure un terzo è stato finora impiegato? Perché? E perché i crediti d'imposta, decisi con legge diversi mesi fa, per determinati tipi d'investimento sono ancora sulla carta, in attesa di non so più quale misura attuativa, fermando opere che sarebbero potute partire da tempo? Diciamoci la verità. Le riforme per spendere meno in tema di pensioni le abbiamo sapute fare; quelle per essere più efficienti e magari, quando è il caso, spendere di più, sono ancora in attesa e, manco a dirlo, noi paghiamo il costo delle riforme non fatte. Nel nostro Paese, come abbiamo visto nei giorni scorsi, investire finisce per essere un azzardo piuttosto che la vocazione essenziale di un imprenditore e, meno che mai, la vocazione essenziale di imprenditori stranieri, che nel nostro Paese cercano di venire il meno possibile. Noi oggi abbiamo la possibilità di recuperare un ritardo. Abbiamo la possibilità di fare presto e fare bene. Nel corso della campagna elettorale ed anche nei mesi scorsi, noi di Scelta Civica per l'Italia ci siamo affannati a ripetere che oggi lo spartiacque fondamentale della politica italiana non è più quello tra la vecchia sinistra e la vecchia destra: il vero discrimine è tra chi vuole cogliere l'occasione offerta dalla crisi per innescare un processo di rapido allineamento dell'Italia ai migliori *standard* europei e chi pensa invece che questo progetto sia velleitario, che il progetto di adeguare l'Italia all'Europa che funziona meglio sia irrealizzabile, perché l'Italia è diversa e perché in Italia queste cose non si possono fare. Noi restiamo dell'opinione che anche in Italia queste cose, e molte altre, si possano fare, e che si possano fare presto e bene.

sono contenta di intervenire dopo che hanno già parlato molti esponenti degli altri partiti. Intervengo anch'io sulla direttiva n. 63 del 2010. Quando ascolto che il traguardo che è stato raggiunto con l'emendamento presentato dal relatore

Eppure la direttiva n. 63 del 2010 detta una nuova disciplina sulla sperimentazione animale: è una normativa su cui io personalmente avanzo critiche pesanti perché, studiando attentamente il testo, ci si rende conto che le sue affermazioni di principio, che possono sembrare condivisibili, sono poi sistematicamente negate da un'infinita serie di eccezioni e deroghe che ne svuotano quasi completamente la portata.

Questo è stato fatto in maniera molto limitata, perché - probabilmente - eravate troppo occupati a distruggere o a lasciar distruggere quanto resta del nostro Stato sociale: avete dimenticato la scadenza e vi siete ricordati di mandare al volo quattro righe per evitare quanto meno le barbarie che prevedevano la sperimentazione su cani e gatti randagi (perché questo è ciò che prevede la direttiva europea che noi stiamo recependo). Allora, Europa comanda e Italia ubbidisce. Ho sentito qui riempirsi la bocca di questa Europa, ma in realtà ciò che facciamo è solamente obbedire a quanto ci viene detto, perché non c'è nessuno di coloro che ci rappresenta che veramente difende i nostri interessi e i nostri punti di vista. vista. Signori, abbiamo imparato a conoscervi. Sappiamo leggere tra le righe e ci sono delle grande falsità nelle affermazioni che fate proprio in base a questo emendamento, che servono solo a mettere una pezza al lassismo in cui questo Paese è ormai costretto a vivere. Infatti, spunta la minaccia dell'infrazione

un vincolo insormontabile quando si parla di difendere i diritti degli animali. Abbiamo presentato tre emendamenti. L'unico che veramente in molti del mio Gruppo vorremmo veder accolto è quello con cui si scelgono la coerenza

riconosce la diversità dell'atteggiamento nei confronti degli animali, collegandola alla differente percezione nazionale (ma noi non siamo più una Nazione), vietando però, poi, ai popoli europei più garantisti, l'esercizio del sacrosanto diritto di poter tutelare veramente i loro amici

18. Avete avuto la compiacenza di leggere gli emendamenti che abbiamo presentato? Se lo aveste fatto, forse avreste notato che erano stati studiati. Essi proponevano procedure volte a garantire, a controllare, a dare trasparenza e serietà e chiedevano solo di evitare ciò che non è scientificamente indispensabile. Non c'era nulla di quel populismo di cui amate riempirvi la bocca per giustificare la nostra esistenza, senza avere il coraggio di riconoscere che ciò è dovuto principalmente al vostro totale fallimento.

ha chiesto di fermarsi un attimo e di poter discutere. Ma era più semplice far finire tutto quanto lì. Noi però abbiamo letto molto bene l'emendamento del relatore che voi avete approvato con grande sollievo. Non vi raccontiamo che cosa dice (anche i colleghi che l'hanno accolto hanno detto che non è poi così rivoluzionario), però vi diciamo che cosa non dice. Non figura assolutamente l'obbligo di sostituire ogni volta in cui sia possibile farlo in modo scientificamente soddisfacente, le metodologie che utilizzano gli animali vivi con quelle che non li utilizzano. Quando non scrivete che c'è un obbligo vuol dire che non obbligate a fare nulla! *(Applausi

È stato vietato esclusivamente l'allevamento dei primati non umani, consentendo il loro libero commercio e la vendita. Quindi, non faremo sperimentazioni su esemplari italiani ma su quelli argentini. È stata eliminata la quota precisa. Non avete mai soldi.

È stata del tutto ignorata la valutazione retrospettiva dei progetti. Vengono permesse le esercitazioni, i corsi sono facoltativi, non c'è l'obbligatorietà di un numero annuo minimo di ispezioni senza preavviso: li avvisiamo e poi facciamo le ispezioni. Obbligo di comunicare annualmente al Ministero le statistiche relative agli animali nati, ceduti, morti. Pubblicazione delle procedure. Partecipazione delle associazioni animaliste. E ci sarebbe tanto altro, ma penso che quanto detto basti e avanzi. Comprendiamo la paura di chi teme che si perda qualsiasi criterio di delega e ancor di più comprendiamo il terrore di chi teme soprattutto coloro che in Italia sono chiamati a prendere le decisioni: voi. Personalmente, accettare questo ennesimo inciucio, giocare al ribasso, al meno peggio, mi induce solo a pensare che purtroppo gli animali non votano e non possono difendersi in questa Assemblea perché non sono considerati altrettanto degni della nostra intelligente e cosciente specie, perché mossi solo dall'istinto e non dalla ragione. E se ragione, però, vuol dire anche buonsenso, se umanità vuol dire non fredda logica ma anche coraggio di saper assumere scelte etiche, allora, a mio avviso, quegli animali sono più umani di coloro che in questa votazione li sacrificheranno, non alla ricerca, ma al libero mercato e al semplice risparmio dei costi aziendali! Lascio quindi alla vostra coscienza stabilire in questa pagina chi sono le vere bestie.

di valori, abbia bisogno di pacatezza, mai come in questo momento, mai come in questo anno in cui una serie di decisioni verranno assunte, una serie di importanti appuntamenti verranno centrati. Ritengo che all'Europa, signor Presidente, guardiamo con fiducia, spesso con circospezione, altre volte con diffidenza. Sono sentimenti che obbligano ad una riflessione. Ci saranno motivazioni, ci sarà un perché tali stati d'animo permeano il contegno delle popolazioni, dei singoli cittadini e delle comunità locali riguardo alla presenza, alla percezione di questa entità straordinaria qual è l'Unione, la vecchia e cara Comunità europea, così come veniva denominata dopo gli albori del famoso MEC, il Mercato comune europeo. Spesso, signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, l'idea di Europa appare distante, scostante. Più volte, nella prassi quotidiana, l'idea che recepiamo dell'entità politica, ordinamentale, economica e finanziaria

il nostro sogno di un continente unito, forte, in grado di giocare la partita della sicurezza e della pace tra i suoi Stati membri e fra le Nazioni del mondo. Ebbene, signor Presidente, attraverso il recepimento della legge di delegazione europea,

che esercitiamo per intero il nostro diritto a criticare l'Europa, ma anche a valorizzarne i punti di straordinaria eccellenza. Siamo convinti che, attraverso questo percorso che qui oggi viene consumato, che è un percorso collettivo, tutti quanti - ognuno per la sua parte, ognuno per la sua cultura e sensibilità politica - potranno dare un contributo straordinario, che a mio parere può può essere ancor più valorizzato se guarderemo insieme all'ideale europeo in termini di opportunità. Con tali sentimenti concludo il mio intervento, sottolineando che questi sono gli impegni che il Parlamento italiano, e il particolare, affida al Governo affinché eserciti per intero la sua capacità di persuasione, ma anche la sua capacità di essere in Europa con grande dignità.

la discussione di oggi sui provvedimenti in votazione è l'occasione per ripensare il rapporto del nostro Paese sia in materia di adempimenti nel quadro della partecipazione all'Unione europea, in particolare relativi alla prevenzione e alla risoluzione delle procedure di infrazione, sia in relazione ai fondi strutturali stanziati in favore del nostro Paese e al loro mancato utilizzo. Ciò anche in relazione all'indiscutibile successo a cui è pervenuto il Governo Letta in merito alla maggiore flessibilità di bilancio a partire dal prossimo anno per i Paesi usciti dalla procedura di *deficit* eccessivo come il nostro, che dimostra come l'assunzione di posizioni determinate e autorevoli nei confronti dell'Europa consente il raggiungimento di traguardi lungimiranti. Il numero relativo di procedure di infrazione a carico dell'Italia, che hanno superato ormai il centinaio, sia per violazione del diritto dell'Unione sia per il mancato recepimento di apposite direttive, deve infatti indurre tutti noi sui tempi e sui modi opportuni di legiferazione delle Assemblee legislative, presi in coerenza con gli indirizzi comunitari e ancor più con una visione chiara ed organica alla quale anche le Regioni devono conformarsi. Al di là di isolate ma sempre più frequenti posizioni antieuropeiste che attraversano talune associazioni in Italia e nel resto d'Europa, è ineludibile un processo di rafforzamento e di integrazione europea, dove l'Italia può

ed è fondamentale, al riguardo, ripensare necessariamente alla gestione dei fondi europei e alla loro spesa celere ed efficiente per garantire sviluppo e occupazione. I dati relativi al ciclo di programmazione europea 2007-2013 indicano una spesa intorno ai 20 miliardi di euro pari al 37,5 per cento, cioè sotto la soglia minima del 40 per cento delle risorse complessivamente assegnate al nostro Paese, che ci pone in una situazione di criticità rispetto alla grave crisi economica che stiamo attraversando e alla costruzione della nuova programmazione comunitaria e regionale che arriverà fino al 2020. In questo momento, dunque, l'Italia contribuisce ai finanziamento dell'Europa ma dai fondi che l'Europa stanzia in nostro favore noi non riusciamo a spendere ed investire opportunamente le somme previste. Dobbiamo dunque prevedere misure di snellimento delle procedure burocratiche che possano accelerare gli interventi, garantendo qualità e selettività della spesa, nonché intervenire sulle Regioni che presentano maggiori ritardi negli investimenti strutturali previsti nelle varie programmazioni territoriali per scongiurare ipotesi di restituzione di risorse e al fine di garantire sviluppo e crescita occupazionale nel quadro dei programmi operativi, nazionali e regionali. Onorevoli colleghi, l'approvazione dei testi oggi in Aula deve essere un primo passo per avviare un percorso nuovo e un più costruttivo rapporto tra Italia ed Europa nel rispetto della reciproca collaborazione e della più incisiva integrazione sociale ed economica. Desidero infine esprimere

Signor Presidente, senatrici e senatori, consentitemi di ringraziarvi per l'interessante discussione che ha avuto oggi luogo in Aula, così come per i proficui lavori che si sono svolti in seno 14a Commissione, per i quali ringrazio i relatori e il presidente Chiti. Credo che il dibattito abbia posto in luce gli elementi essenziali dei testi che oggi ci sono sottoposti, in particolare dei due testi legislativi: da una parte, questi testi consentiranno alla fine consentiranno alla fine dell'intero *iter* legislativo parlamentare - ma consentono nell'ambito dell'attuale discussione - di dare piena attuazione agli impegni assunti dal nostro Paese in seno alla partecipazione democratica al processo legislativo ed istituzionale dell'Unione europea; dall'altra parte, questo permette anche di individuare una serie di snodi importanti che stanno per essere introdotti e potranno essere introdotti nel nostro ordinamento sulla base della legislazione che abbiamo contribuito ad adottare nell'ambito dell'Unione europea. È stato evocato da più intervenienti il recupero di un ritardo; un ritardo che si era effettivamente accumulato nel corso degli ultimi anni a causa della mancata possibilità di portare a termine l'*iter* legislativo relativo alle due leggi comunitarie del 2011 e del 2012. Questo ritardo si innestava, purtroppo, su un precedente ritardo che aveva caratterizzato l'*iter* legislativo della legge comunitaria del 2010.

scaturiscono da meccanismi istituzionali a livello di Unione europea rispetto ai quali il nostro Paese è pienamente partecipe: è partecipe perché, in seno al ramo legislativo - Consiglio, partecipano, per le varie tematiche, i Ministri del nostro Governo ed è partecipe perché, in seno al ramo legislativo - Parlamento europeo, partecipano i membri eletti a suffragio universale in Italia. Si tratta, quindi, di norme che non provengono da un luogo metafisico, come Europa o Bruxelles, ma che scaturiscono da discussioni politiche e democratiche che si svolgono in seno a un Parlamento eletto a suffragio universale e in seno a un Consiglio ove partecipano Ministri individuati attraverso procedure democratiche a livello dei vari Paesi. Il vero problema, quindi, non sta nella fase a volte (o spesso) travagliata, discendente, di recepimento, quella che noi ora stiamo vivendo, ma nella preparazione e nella attenzione alla fase ascendente, quella in cui, in sede di Unione europea, si formano le norme. A questo proposito, la legge n. 234 del dicembre 2012, che ha innovato la precedente legislazione, ha reso il Parlamento molto più centrale e molto più coinvolto nella partecipazione alla cosiddetta fase ascendente, quella in cui - lo ripeto - i Ministri del Governo partecipano in seno al Consiglio dell'Unione europea alla discussione e all'adozione delle direttive che, successivamente, devono essere recepite. Come sapete, le Commissioni parlamentari hanno la possibilità di convocare i Ministri prima che questi partecipino ai Consigli in sede di Unione europea e possono sentirli successivamente per comprendere cosa è accaduto e dare, naturalmente, linee d'indirizzo. Credo sia una facoltà molto importante che è lasciata al Parlamento. Ripeto: è nella fase di elaborazione e di adozione delle norme in sede europea che dovrebbero essere poste tutte quelle questioni di specifica rilevanza per gli ordinamenti nazionali che poi dovranno recepire queste norme, in maniera che esse siano tenute presenti o, eventualmente, non presenti, ma sempre tramite un procedimento di democrazia. Scoprire i problemi legati alla legislazione europea quando questa è stata adottata e deve essere discussa per il recepimento ‑ certamente con margini di manovra, ma comunque limitati ‑ è tardi. Scoprirli addirittura dopo il recepimento, come sovente accade, è ancora più tardi. La partecipazione democratica e la tutela degli interessi del Paese e dei cittadini si svolgono attraverso la fase ascendente e - lo ripeto - attraverso il controllo che il Parlamento può esercitare - con lo strumento rafforzato della citata legge n. 234 - sul Governo quando partecipa alla fase legislativa in sede europea, oltre che attraverso i contatti che il Parlamento può e, a mio modesto parere, dovrebbe mantenere con i membri italiani del Parlamento europeo, per assicurare una dinamica di cinghia di trasmissione funzionale.

La legge n. 234 però, ancora una volta, viene incontro all'esigenza di trattare su corsie specifiche provvedimenti europei di particolare rilievo o complessità: altra facoltà che risiede nelle mani del Parlamento. Quindi, potrà essere opportuno, anche per motivi di economia dei lavori parlamentari, raggruppare negli strumenti legislativi della legge europea e della legge di delegazione europea le varie disposizioni e gli atti di attuazione, ma per le situazioni più articolate e complesse possono essere identificati dei veicoli *ad hoc* e chieste dal Parlamento delle sedi di dibattito *ad hoc.* È una facoltà di cui penso potrete fare uso quando lo riterrete opportuno. Certamente l'adozione delle disposizioni contenute nei due strumenti legislativi oggi sottoposti al vostro voto e al vostro dibattito permetterà di chiudere un numero importante di procedure di infrazione alle norme europee (all'incirca una ventina, per essere precisi), oltre che scongiurarne altre che sarebbero scattate o che scatterebbero qualora non fossero adottati i provvedimenti. Vi ricordo - ma, certamente che l'Italia è il Paese che ha il maggior numero di procedure di infrazione. Non si tratta - lo ricordo ancora una volta - di dissensi filosofici: sono procedure concrete che determinano situazioni di illegalità per il nostro Paese

prima della Comunità europea, che è stata ricordata, poi successivamente dell'Unione europea. Non si tratta, quindi, ancora una volta di imposizioni esogene, ma partecipazione a sistemi ai quali democraticamente e liberamente aderiamo. È evidente che ritardi nell'attuazione della legislazione, infrazioni, ritardi nell'utilizzo dei fondi europei e nella spesa determinano una complessiva riduzione dell'affidabilità e di quella tante volte nominata credibilità del nostro Paese nelle sedi europee. Se vogliamo che realmente l'Italia, a prescindere dai Governi e dai Ministri,

Muoversi nell'ambito delle regole significa non accettare supinamente altre regole, ma avere, al contrario, la possibilità di discutere, di compartecipare e di influire sull'adozione delle regole e delle linee politiche di indirizzo. Qualcuno di voi ha voluto ricordare l'importanza di quanto abbiamo nuovamente focalizzato ieri a seguito delle dichiarazioni del Presidente della Commissione europea, che altro non facevano che dare seguito operativo alle decisioni prese dal Consiglio europeo, peraltro reiterate più volte (la prima volta nel dicembre del 2012, una seconda volta nel marzo del 2013, una terza volta nel giugno del 2013), vale a dire quella flessibilità consentita dalle norme, pur rigorose, sulla salute dei conti pubblici che consente di fare investimenti pubblici produttivi, soprattutto durante questo periodo di crescita. che questo risultato importante fatto proprio dai capi di Stato e di Governo è stato notevolmente stimolato dall'iniziativa italiana. Così come fu su iniziativa italiana che nel febbraio del 2012 si iniziò a parlare di crescita e di occupazione a livello europeo. Così come è stato grazie a un forte stimolo d'iniziativa italiana che nel Consiglio europeo della settimana scorsa sono stati incrementati i fondi a disposizione per la lotta contro la piaga della disoccupazione giovanile. Ci si può quindi far valere a livello

con le carte in regola in merito agli adempimenti. Credo che con il passo che stiamo per compiere con l'esame parlamentare dei due disegni di legge ci stiamo avviando nettamente in quella direzione per quanto riguarda i recepimenti legislativi. Di questo ringrazio ancora una volta il Senato.

indicata come proposta n. 3. Il Governo tiene peraltro a dichiarare che molti, per non dire la grande maggioranza, degli aspetti contenuti nelle altre due proposte di risoluzione lo trovano consenziente.

1a Commissione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge n. 588, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza i seguenti pareri: sull'emendamento 26.200 parere non ostativo, a condizione che: a) al comma 2, il parere dell'ISPRA, ivi previsto, non abbia carattere vincolante; b) al comma 4, sia soppressa la previsione del versamento di una tassa regionale per l'esercizio della deroga, in quanto lesiva dell'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni; c) al comma 5, sia soppresso il secondo periodo, dal momento che la norma ivi prevista attribuisce alla Regione competenze riservate, in via esclusiva, allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; d) sia soppresso il comma 6, in quanto appare più ragionevole - e compatibile con i rispettivi ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni la procedura prevista all'articolo 26, comma 2, capoverso "Art. 19-*bis*", comma 4, del testo; - sugli emendamenti 26.201 e 26.100 parere non ostativo, a condizione che il parere dell'ISPRA ivi previsto, non abbia carattere vincolante; - sui restanti emendamenti parere non ostativo».

presupposti: - che, quanto all'articolo 1, comma 4, l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 per la copertura di spese non previste dalla legislazione vigente, e comunque nei soli limiti delle necessità connesse all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, abbia carattere eccezionale e riguardi in ogni caso un numero limitato di direttive tra quelle oggetto di recepimento; - che, rispetto all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, si possa provvedere al potenziamento dell'attività ispettiva con le risorse previste a legislazione vigente; che, quanto all'articolo 8, esso consenta l'abrogazione di norme non più applicate in ragione della loro incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che pertanto non vi siano effetti negativi sulle entrate; che, rispetto all'articolo 11, i possibili maggiori costi gravanti sulla Banca d'Italia e sulla CONSOB possano essere integralmente finanziati a carico dei soggetti vigilati tramite le rispettive contribuzioni; - che il recepimento della direttiva 2011/95/UE non comporti un ampliamento della platea degli aventi diritto allo *status* di rifugiato, e che gli eventuali maggiori costi derivanti dall'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva saranno oggetto di puntuale individuazione nell'ambito dello schema di decreto legislativo di recepimento; che, quanto alla direttiva 2011/99/UE, l'applicazione del criterio di riparto delle spese tra Stato di emissione dell'ordine di protezione e Stato di esecuzione, previsto dalla direttiva medesima, non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; - che, rispetto alla direttiva 2012/18/UE, l'attività ispettiva ordinaria sarà finanziata a carico dei gestori degli impianti, mentre quella di tipo straordinario potrà essere svolta a risorse invariate; - che, quanto alla direttiva 2012/34/UE, l'obbligo di garantire l'equilibrio finanziario del gestore dell'infrastruttura ferroviaria (articolo 8, comma 4) non si possa tradurre in un aggravio per l'erario. Il parere è invece di contrarietà sull'articolo 4, comma 1, e sull'articolo 5. In merito all'articolo 12 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 1, lettere *a)*, *l)* ed *m)*, mentre, sulla parte restante dell'articolo, il parere è di contrarietà. Il parere è reso, è reso, altresì, con la seguente osservazione: quanto alla direttiva 2012/52/UE, essendovi la necessità di garantire la neutralità finanziaria del riconoscimento delle ricette mediche in ambito europeo rispetto agli obblighi di rimborso del costo dei medicinali a carico del Sistema sanitario nazionale, appare indispensabile che l'invarianza degli oneri venga confermata da parte della competente Amministrazione prima della conclusione dell'*iter* del provvedimento presso questo ramo del Parlamento. In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.101 e Sull'emendamento 3.0.3 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 12.100, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma

Commissione di merito ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che: - l'articolo 8 - che amplia i casi di esenzione dall'imposta di stazionamento per gli aeromobili privati - comporti un decremento di gettito di trascurabile entità; il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie rechi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'articolo 13, comma 2, lettera *a)*; - le modifiche alla disciplina sul monitoraggio fiscale contenute nell'articolo 9 -ed in particolare il comma 1, lettera capoverso "Art. 4", comma 2, che introduce una ritenuta d'acconto del venti per cento sui redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria - non comportino un decremento di gettito, rispetto alla normativa vigente. Il parere è altresì reso con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 24,

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie non appare del tutto conforme ai principi contabili vigenti; - la copertura di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *c)*, assorbendo quasi la metà dello stanziamento iscritto, a partire dal 2014, sul Fondo nazionale per le politiche sociali, espone al rischio di ridimensionare ulteriori interventi finanziati dal medesimo Fondo; - il ricorso, disposto dai medesimo articolo 13, comma 2, lettera *d)*, a quota parte dell'otto per mille IRPEF di spettanza statale, rappresenta il perpetuarsi di una prassi basata sul ricorso a tali stanziamenti per finalità difformi rispetto alla legge istitutiva del meccanismo dell'otto per mille; - l'articolo 30 - che consente l'istituzione di ulteriori sezioni presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale - reca un onere coperto sul bilancio a valere su risorse che dovrebbero risultare interamente impegnate legislazione vigente. Per quanto attiene agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 26.200 (già 27.1), 26.204 (già 27.10), 33.200

e l'analogo 34.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti». i disegni di legge e sulla proposta di risoluzione n. 3, accettata dal Governo, avrà luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 587,

(testo 2) ha lo scopo di impegnare il Governo, nel concedere la delega, a rivedere le tariffe elettriche per renderle più adeguate a un mercato aperto.

e un adeguamento delle tariffe elettriche più congruo al mercato certamente andrà in direzione di spingere all'utilizzo di questo tipo di strumenti.

sostanzialmente una condizione *ex* articolo 81

In merito, invece, agli emendamenti 12.100 e 12.101, in ossequio al lavoro svolto in Commissione e all'equilibrio raggiunto, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore,

almeno si consenta, con l'emendamento approvato, ai veterinari di poter lavorare sugli animali, cosa che nel testo originario non era prevista. Sono però assolutamente in

articolo, che delega il Governo rifacendosi alla normativa europea, consentirà all'Italia di fare tutte quelle cose che nella prima parte dell'articolo noi vogliamo, in maniera improvvida, vietare. Per fortuna, ci sono normative europee ed internazionali e con

tutte le istanze, etiche e morali, compresa la possibilità di vietare gli xenotrapianti di organi, ma non di parti di esse. Stupisce che ancora qualcuno abbia dei dubbi sulle valvole dei maiali.

entrare adesso nelle sale di cardiochirurgia e a quantificare quante siano le valvole biologiche attualmente in uso. Le valvole biologiche, come sapete tutti, oltre a dare problemi di rigetto, infezioni e endocarditi, hanno anche un altro inconveniente: non

lo stesso esempio da lei riferito in Aula, onorevole Giovanardi, ovvero il talidomide, è infatti alla storia il fatto che tale medicinale non abbia prodotto bambini focomelici perché non sufficientemente sperimentato sugli animali. Infatti, dopo tre anni di prove sugli animali, la «Chemie Grünenthal» lo mise in commercio come innocuo tranquillante adatto soprattutto alle gestanti, autorizzandone la libera vendita senza alcuna prescrizione medica in tutta la Germania, con lo slogan: «Innocuo come una zolletta di zucchero». Solo Solo dopo la catastrofe teratologica che procurò la nascita di 10.000 bambini focomelici nel mondo si decise di sperimentare in modo massiccio, ovvero a dosi altissime su oltre 150 diverse razze di conigli, e si ottennero solo alcuni nati focomelici, il che dà alla vicenda un senso completamente diverso, come è ben comprensibile a chiunque faccia della ricerca seria e coerente. Occorre anche evidenziare che se i se i farmaci dovessero essere sperimentati su un elevato numero di animali sarebbero tutti ritirati dal commercio, perché qualsiasi farmaco, ad oggi, ha degli effetti collaterali negativi su almeno una specie animale. Ricordo inoltre in questo contesto che noi non avremmo farmaci come l'aspirina, noto a tutti e universalmente utilizzato, se l'avessimo sperimentato soltanto sugli animali. Ci tengo a rimarcare che il Movimento 5 Stelle in queste dichiarazioni di voto, a

Grazie e non frutto di stampa, *gossip* o quant'altro. Il Movimento 5 Stelle ha fatto un voto etico, è vero, perché vorrebbe che l'Italia

però oggi devo dire che mi associo totalmente alle sue posizioni e alle sue preoccupazioni.

perché altrimenti ci metteremmo in una situazione di carenza, di *deficit* e di incapacità a competere con il resto del sistema economico Quindi non è questione soltanto di voler essere animalista o non animalista (credo di essere un animalista convinto, in quanto in famiglia mantengo alcune decine di animali), però il però il problema è: la sperimentazione, se non si fa sugli animali, su cosa si fa? La sperimentazione necessaria: non le degenerazioni, ma quella necessaria, quella indispensabile. La sperimentazione, se non si fa sugli animali, finisce per essere fatta sugli uomini. Questo è il punto. Chiedo allora il rispetto rigoroso della direttiva europea una richiesta pressante al Governo affinché nei suoi provvedimenti non si distacchi dalla direttiva europea.

Su tutte le disquisizioni scientifiche vorrei dire soltanto una cosa, molto chiara: ogni specie è unica, il modello animale non è

a questa riflessione per dire che mi asterrò dalla votazione, a differenza del mio Gruppo, ma voglio fare una riflessione ad alta voce, affinché tutti i colleghi che sono presenti in quest'Aula possano prendere effettivamente coscienza delle parole che noi utilizziamo.

l'ordine del giorno G100 per estraneità al contenuto del disegno di legge in

Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.100 volevo evidenziare che esso è un necessario chiarimento all'emendamento già votato dalla Commissione perché i cittadini extracomunitari devono chiaramente essere parificati ai cittadini italiani.

sottostare agli stessi principi dei cittadini italiani. Non vogliamo discriminare nessuno, però pari trattamento. Pertanto invito il Governo

Il ministro Moavero mi pare che confermi quell'opinione. Poi la questione potrà essere oggetto in altri momenti di approfondimento. Ne capisco l'importanza, certamente.

la possibilità che qualcuno di noi, perché parlo anche a nome degli altri Gruppi, abbia il desiderio, comunque nell'esercizio di un suo diritto, legittimo, mi sembra, di chiedere il voto elettronico, siamo in un altro Paese.

Questa procedura d'infrazione riguarda le rappresentanze sindacali nelle aziende. Purtroppo, però, questo atto del Senato non contiene la procedura d'infrazione 2010/2124 relativa alla stessa direttiva europea, che invece riguarda sottolineo l'abuso, non l'uso - che fa l'Italia dei contratti a tempo determinato del personale della scuola ATA e docenti. Data l'importanza che il settore dell'istruzione deve avere per questa Assemblea e per l'operato del Governo, ritengo importante porre all'attenzione questa questa ulteriore procedura d'infrazione, che non solo è allo stadio della messa in mora complementare, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma addirittura è oggetto di svariati ricorsi che gli insegnanti precari hanno posto in essere, molti dei quali giunti già a sentenza di primo grado favorevole agli insegnanti stessi.

Questo proprio per venire incontro a quegli insegnanti che, anziché essere tutelati e valorizzati nel loro importantissimo ruolo, vedono i loro diritti loro diritti calpestati e sono quindi costretti a ricorrere contro lo Stato per vederne il riconoscimento. Auspico pertanto che il Governo accolga questo importantissimo ordine del giorno relativo al settore della scuola

- ho votato a favore - però onestamente non ne conosciamo né la riformulazione, né la discussione che si è svolta. Credo che sarebbe molto più corretto

*(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante dispositivo elettronico.

con l'articolo 20 si va a recepire le direttive sullo smaltimento dei rifiuti delle imprese estrattive. Io provengo da Carrara e quindi

l'adozione di criteri uniformi tali da garantire la piena sostenibilità ambientale degli interventi estrattivi. Quando si lavora in cava i danni i danni ambientali sono immensi: si va non solo a deturpare il paesaggio ma anche a rovesciare

estrattivo; le cave di Livorno, sulle colline di Campiglia Marittima e San Vincenzo,

quando viene dismessa, spesso diventa una discarica a cielo aperto. Nel Comune di Massa, l'ex cava Viti ormai è una discarica che da abusiva è diventata quasi legale senza che nessuno faccia nulla. Questo è quello che hanno fatto i politici italiani sul nostro territorio. Inoltre, per i rapporti che si sono stabiliti nel corso degli anni tra gli imprenditori locali e le amministrazioni che si sono susseguite, devono essere revisionati, secondo un criterio univoco su tutto il territorio. Alcune Regioni legiferano sull'azione estrattiva,

per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; le lettere *g)*, *h)* ed *i)* del comma 1 dell'articolo 21 riscrivono i primi due commi

sulla partecipazione del pubblico al procedimento autorizzatorio relativo ai depositi dei rifiuti di estrazione, prevedendo adeguate forme di pubblicità; impegna il Governo: a valutare l'opportunità di garantire una piena e trasparente informazione sui procedimenti autorizzatori relativi ai depositi dei rifiuti di estrazione a tutti i cittadini che vivono nei territori coinvolti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, anche attraverso la pubblicazione della documentazione informativa su tutti i quotidiani a diffusione sia regionale che provinciale.

Signor Presidente, chiedo una precisazione rispetto alla ripresa dei nostri lavori.

l'articolo 28 risolve lo stesso problema.

Dichiaro aperta la votazione.

funziona molto bene e dal punto di vista scientifico è quanto di più serio si possa immaginare. Non vedo per quale motivo dobbiamo togliere questa possibilità. Chiedo

Dichiaro aperta la votazione.

«Disposizioni di attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche ed Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009».

e buon lavoro, visto che il pranzo è saltato.